Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi il Senato si avvia ad approvare una nuova e diversa disciplina del condominio

Quella condominiale è una materia complessa, sia sotto il profilo giuridico, per le sue diverse implicazioni, sia soprattutto sotto quello della quotidianità degli eventi che a questa materia si riferiscono. Se le stime sono prossime alla realtà (e lo sono), almeno 12 milioni di famiglie - circa 40 milioni di persone - sono interessate nella loro vita quotidiana da piccoli e grandi problemi, che hanno investito l'autorità giudiziaria con una mole di ricorsi e complessivamente di contenzioso, che evidentemente una riforma di sistema dovrebbe cercare di evitare.

sia per la difficoltà di ricomprendere in una disciplina accurata fattispecie disparate e di difficile riconduzione a norme astratte che possano valere *erga omnes*, per materie che poi si esplicano con una miriade di casi. Questa riforma era stata prospettata come un intervento chirurgico, finalizzato ad aggiornare una secolare disciplina sul condominio

Per esempio, nonostante sia stato bocciato in Commissione, e ieri anche in Aula, l'emendamento che riconosce capacità giuridica al condominio, di fatto è stata introdotta una modifica una modifica importante: il condominio da semplice soggetto aggregativo nel quale i condomini definiscono come gestire le parti comuni dell'edificio e individuano i criteri per la ripartizione delle spese

non dovesse riguardare il trasferimento o la costituzione di diritti reali, di fatto riconosce al condominio una soggettività che prima non aveva.

dovrebbe rispondere con il suo patrimonio, che continua a rimanere del tutto differente da quello dei condomini, e solo in via sussidiaria dovrebbero rispondere coloro che per il condominio hanno agito, ossia gli amministratori, ovvero chi ha autorizzato - i condomini consenzienti - le operazioni soggette a trascrizione. C'è uno sforzo per dare importanza e rilevanza alla figura professionale degli amministratori, con l'introduzione del rendiconto.

assicurazione particolare ma una garanzia fideiussoria calibrata sull'ammontare degli oneri condominiali previsti, garanzia che di fatto è fortemente vessatoria nei confronti della categoria degli amministratori, e che poteva essere parametrata in maniera diversa. Mi auguro che, su detto nonché su quelli che ho precedentemente illustrato, l'altro ramo del Parlamento possa apportare quelle modifiche che noi non siamo riusciti insieme ad individuare. Mentre la norma, coerentemente, cerca di ridurre il *quorum* per determinate categorie di deliberazione, di colpo reintroduce - avevo già sollevato la questione ieri in Aula - l'unanimità per la modificazione delle tabelle millesimali. Questa è stata una *vexata* *quaestio* nel corso degli anni, finalmente risolta anche in maniera pregevole dalle sezioni unite della Cassazione, che avevano spiegato perché

davanti all'autorità giudiziaria solo perché si rifiuta una modifica di tabella millesimale, instaurando così un contenzioso. Noi riteniamo che la materia sia stata migliorata per un verso, che per altro verso sarebbe stata, e sia, meritevole di ulteriori e puntuali approfondimenti. Per queste ragioni, l'Italia dei Valori, che apprezza il lavoro complessivamente svolto, svolto, si asterrà su questo disegno di legge, e si augura che nel corso dell'*iter* parlamentare si possano apportare quelle correzioni che rendano la materia regolata più fluida e soprattutto più fruibile nei confronti delle decine di milioni di italiani coinvolti in questioni che col condominio hanno a che fare.

Ma tant'è: ancora una volta si è voluto mettere mano ad una riforma per far passare all'esterno un messaggio un messaggio di innovazione. Credo che questa normativa sia tutt'altro che ambiziosa, che sia assolutamente di basso profilo e comporti maggiori oneri per i condomini. Il nostro impegno, sin dall'esame in Commissione, è stato orientato *in primis* a tutelare il cittadino - soprattutto il piccolo proprietario - salvaguardandolo dall'eventuale rincaro dei costi di gestione conseguenti alle modifiche che si vogliono introdurre.

preannunciato un voto assolutamente negativo a questa norma, ma tale disponibilità ci ha indotto a modificare

il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo disegno di legge, frutto di un lavoro meticoloso, lungo, svolto prima dal Comitato ristretto costituito in seno alla Commissione giustizia e poi dalla Commissione Il lavoro è stato svolto in contatto e confronto diretto con autorevoli esperti della materia condominiale; una materia molto difficile, tecnicamente molto complessa ma che riguarda la gran parte dei cittadini di questo Paese. Abbiamo già detto ieri che il riordino della disciplina del condominio negli edifici, regolamentata dal codice civile del 1942, era un'esigenza avvertita da anni alla luce del cambiamento radicale dei modelli di insediamento abitativo. oggi se un cittadino italiano vuole capire quali sono le norme che disciplinano il condominio deve non solo rifarsi alle poche norme del codice civile del 1942, ma ai numerosi repertori della giurisprudenza di merito e di legittimità, alle numerose sentenze di Cassazione e dei tribunali intervenute sulle norme del codice civile. Quindi, occorre uno sforzo interpretativo notevole per riuscire a comprendere il senso di quelle norme del codice civile, sforzo interpretativo reso necessario dai settant'anni che sono passati dall'emanazione di quelle norme. Tale sforzo comporta anche un notevole contenzioso, che sta congestionando i nostri tribunali; credo che la materia condominiale sia una delle materie maggiormente trattate nelle aule giudiziarie, intasando gli uffici giudiziari.

Sui punti qualificanti mi rimetto agli interventi di ieri, soprattutto quello del relatore Mugnai, che ha chiarito esemplarmente i punti importanti di questa riforma. A me interessa indicarne due in particolare, che riguardano la figura dell'amministratore di condominio. Oggi per fare l'amministratore di un condominio l'unico requisito richiesto è quello di avere 18 anni.

Non è un caso che questa riforma preveda un registro pubblico degli amministratori condominiali, custodito presso le Camere di commercio, e che tipicizzi i comportamenti che portano alla revoca dell'amministratore incapace. Gli amministratori condominiali - non dobbiamo dimenticarlo - movimentano ogni anno più di 15 miliardi di euro, dunque sono uno snodo essenziale anche del circuito economico. Ecco perché questa riforma ha voluto fortemente una polizza

approvata non si sarebbe verificata la vicenda della fuga con la cassa di un amministratore condominiale milanese che ha lasciato pochi mesi fa 8 milioni di euro di debiti, tra fornitori non pagati e tasse condominiali evase.

credo che già questo sia un risultato importante. Quindi, maggiore responsabilizzazione dell'amministratore condominiale e maggiore trasparenza nella contabilità e nella gestione condominiale. Certo, le risposte di ingegneria giuridica alle esigenze sociali avvertite potevano anche essere diverse. Ieri, si è parlato a lungo della capacità giuridica, ma crediamo che la riforma che oggi approviamo sia una buona riforma

riforma con il relatore Mugnai, leggere un comunicato stampa di un'importante associazione di categoria come la Confedilizia, che ieri parlava di una riforma di basso profilo, fatta in un clima conciliare di altri tempi. Crediamo che il metodo di lavoro scelto dalla Commissione giustizia possa costituire invece un modello virtuoso, sia sotto il profilo della tecnica legislativa che dei risultati ottenuti. Quest'Aula ha licenziato poche settimane fa attraverso quel metodo di lavoro la riforma della professione forense, che attendeva da settant'anni di essere approvata; oggi, dopo altri settant'anni di attesa, approviamo finalmente la riforma del condominio.

approdato in Aula e che oggi siamo chiamati a votare costituisce il punto di arrivo, come ha fatto rilevare anche il relatore ieri, di un confronto che si è sviluppato nel corso di tre legislature. Sia quello che abbiamo presentato come Gruppo del Partito Democratico che gli altri disegni di legge rappresentano, con alcune varianti, il risultato del confronto che si è sviluppato nella Commissione giustizia nelle due legislature precedenti su testi che sono poi confluiti in quello elaborato dal Comitato ristretto e dalla Commissione giustizia, unitamente ad un consistente numero di emendamenti del nostro e di altri Gruppi parlamentari. Non era facile pervenire ad un testo condiviso e soprattutto non era semplice rappresentare in esso le molteplici problematiche sottese alle esigenze della riforma, da anni invocata da soggetti associativi e professionali e da molti cittadini attenti all'evoluzione di questa materia. Se si è riusciti, pur con punti di vista che sono rimasti diversi su alcune proposte emendative, a definire il testo che oggi licenziamo in prima lettura è stato grazie al lavoro approfondito e prolungato di molti colleghi, e di ciò voglio dare atto al relatore e al sottosegretario Alberti Casellati, così come ai colleghi del nostro e degli altri Gruppi, a partire dal collega Guido Galperti, che ha lavorato molto a questo testo e che voglio ringraziare insieme a tutti gli altri che hanno mostrato impegno e dedizione. Non era facile, perché questa materia, più di altre, ha visto ampliare costantemente nel corso degli ultimi settant'anni la platea degli interessati (da una minoranza di cittadini interessata alla materia del condominio si è passati ad una larghissima maggioranza

come e più che in altri settori sociali e economici, ha dovuto supplire alla pigrizia e all'inerzia del legislatore in questi decenni.

dell'incertezza normativa e quindi dei diritti e dei doveri di ciascuno. È stato il metro delle virtù, dell'inventiva, del progresso dei cittadini italiani e, al contempo, dei loro vizi, quelli della litigiosità appunto e, a volte, dell'egoismo, a discapito di relazioni sociali più serene e corrette. Se la domanda è dunque volta a capire se serviva un intervento di riforma profondo, di riscrittura del *corpus* di norme codicistiche, invecchiate e mutilate dai mille interventi di interpretazione evolutiva e creativa della giurisprudenza, allora la risposta non può che essere affermativa: sì, serviva, serve una seria riforma del condominio. Se invece ci poniamo un'altra domanda, e cioè se questa è la migliore delle riforme possibili, quella che riconcilia le norme giuridiche con la continua evoluzione delle innovazioni tecnologiche, dei costumi, dei servizi che ruotano attorno alla casa in condominio la risposta è meno netta: non è la migliore riforma possibile; è semplicemente la riforma possibile, quella che in questo ramo del Parlamento si è riusciti, con largo confronto e consenso, a definire. La dimostrazione che questo è il giudizio più equilibrato la possiamo ricavare proprio dall'esame dei residui emendamenti esaminati in Aula ieri, dopo che molti emendamenti nostri e di altri Gruppi sono stati approvati in Commissione. alle proposte di introduzione nell'ordinamento della capacità giuridica del condominio (di cui abbiamo parlato ieri, appunto) e delle norme sulla semplificazione e accelerazione della possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle parti comuni degli edifici, norme da noi proposte e non approvate, che avrebbero segnato ulteriormente in senso positivo il contenuto della riforma. Purtuttavia, vi è uno sforzo di adeguamento ai cambiamenti che in questi decenni si sono prodotti nella vita e nel funzionamento dei condomini, ed è stato positivamente valutato dal nostro Gruppo, a partire dal lavoro svolto in Commissione. questo testo recepisce largamente i contenuti del nostro disegno di legge, il primo che è stato presentato, sia in questa che nelle precedenti legislature,

alla possibilità di disporre in modo più agevole delle parti comuni che hanno perso la loro destinazione, all'introduzione della nozione di condominio orizzontale. E poi, le nuove norme che rendono più agevoli gli interventi di utilità sociale (quali quelle in materia di sicurezza e salubrità degli edifici), quelle relative alle barriere architettoniche, al risparmio energetico (compresa la problematica antica del distacco dagli impianti di riscaldamento centralizzati), agli impianti tecnologici (compresi quelli destinati alla ricezione radiotelevisiva), alla realizzazione dei parcheggi nei condomini; il complesso di norme sulla nomina e revoca, sugli obblighi, sulla responsabilità e sulle garanzie par l'amministratore del condominio, con l'introduzione di un registro pubblico degli amministratori; la rivisitazione del funzionamento delle maggioranze assembleari, del sistema delle impugnazioni, del realizzo dei crediti nei confronti dei condomini, e diverse altre norme positive che, così come altre norme, avranno bisogno di una verifica più attenta in seconda lettura, certo - concreta, sul campo, per verificarne l'efficacia. Dunque, questo testo, che certo non è il migliore possibile - come dicevo - e che mi auguro venga ulteriormente vagliato in seconda lettura, costituisce un significativo passo avanti rispetto alla disciplina oggi vigente. Una forza autenticamente riformista come la nostra, che si è fatta carico prima di altri di presentare una proposta e di migliorarla, non può pertanto, con le riserve e gli auspici che abbiamo formulato, sia in Commissione che qui in Aula, che esprimersi in senso positivo all'approvazione di questa importante riforma. Quando si affrontano temi che riguardano la vita dei cittadini il Partito Democratico c'è, con le sue proposte e con l'attitudine al confronto costruttivo. Purtroppo, pochissime sono state le occasioni offerte in questa legislatura caratterizzata dalla chiusura del Governo e della maggioranza al confronto, da decreti e voti di fiducia come mai prima si era verificato. Questa è una delle pochissime riforme elaborate dal Parlamento in piena autonomia, e noi ne siamo stati

in sede di dichiarazione di voto si deve manifestare un giudizio di sintesi, avendo rimesso alla discussione e alla trattazione degli emendamenti i singoli problemi affrontati. Avendo anche ascoltato le dichiarazioni di voto degli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, sono confortato nell'affermare che, al di là dei molti distinguo, dobbiamo darci atto reciprocamente che si tratta di una buona legge. È una buona legge, il buon risultato di un percorso lungo, svolto praticamente da tutti i membri della Commissione giustizia del Senato, coordinati dall'eccellente lavoro del senatore Mugnai, che va sinceramente ringraziato in questa sede. del Popolo della Libertà ha contribuito con tre proposte di legge: quella del senatore Pastore e di altri senatori, quella dello stesso senatore Mugnai, quella del senatore Carrara e di altri Si è arrivati ad un testo che ci permette, come altri hanno anche riconosciuto dai banchi dell'opposizione, un cospicuo e concreto passo in avanti rispetto a quella che era la normativa riveniente essenzialmente dal codice civile del 1942. In quell'epoca il legislatore, anche in quell'occasione - debbo dire - equilibrato e lucido,

robusta e coerente, rapportata al suo tempo naturalmente, e fece quella scelta che anche in altri passi ha fatto, cioè di entrare nello specifico di una normativa ma dando anche per assunti, per acquisiti alla cultura giuridica concetti e nozioni sui quali non si è intrattenuto filosoficamente, riportandosi alla nozione dei fatti, degli avvenimenti, delle consistenze patrimoniali come vigevano ed erano in essere nel sentire comune, nel patrimonio dei concetti diffusi.

di straordinaria manutenzione, se posso esprimermi così riguardo alla normativa relativa al condominio. D'altra parte, onorevoli senatori, non è che ogni riforma debba essere una rivoluzione: può essere anche una riforma che mantiene alcuni concetti portanti, fondamentali, ma incide sull'articolazione delle normative per il buon funzionamento di un fenomeno complesso com'è il condominio, fenomeno che - lo sappiamo tutti - si è trasformato nel corso dei decenni, perché si è trasformata ontologicamente la comproprietà, il modo di possedere i beni, di farne uso, di metterli a frutto, di trasferirli e di amministrarli per il comune e per il singolo interesse. si tratta di un insieme di norme non tutte coerenti: io invece vedo che vi è una coerenza che lega questo insieme di norme. Si è detto che forse si innescheranno nuovi costi a carico dei condomini: questo non mi sento di escluderlo, per il semplice fatto che la nostra società oggigiorno impone tante di quelle regole, tante di quelle procedure, tanti di quegli accorgimenti e servizi aggiuntivi che fatalmente non possono

ringrazio, onorevole Presidente. Si parlava di maggiori costi: ebbene, questo non mi sento di escluderlo, perché - ripeto - i servizi, le sicurezze, il di più che si richiede oggi nella nostra società fatalmente talvolta dà luogo a costi. D'altra parte, siamo molto strani, non solo come legislatori ma come società, in quanto per un verso chiediamo semplificazione, meno norme, sfrondamento di norme, e un minuto dopo chiediamo più norme, più interventi, più disciplina dei fenomeni nuovi che si verificano nella società. Dunque, anche per il condominio, che - ripeto - il legislatore il legislatore del '42 ha normato con una semplicità e una complessità parametrate al suo tempo, oggi vogliamo delle normative che ci tutelino di più sul piano della sicurezza,

che oggi non attengono più soltanto all'amministrare nel senso corrente del termine (fare la minuta riparazione degli impianti che si rompono, curare l'igiene, la pulizia delle scale), ma comportano tutta una serie di denunzie, scadenze, esposti: tutta una serie di servizi, anche di carattere burocratico, che nessuno dei condomini vuole più assumere su di sé. Questo comporta necessariamente anche una ridefinizione e un arricchimento della normativa che disciplina

colui che si trova ad amministrare. Pertanto, rispetto a tutti questi modi d'essere nuovi, è chiaro che si richiede una normativa più complessa, talvolta più sofisticata, ed è quello che è stato fatto con lo sforzo lodevole di impegno portato oggi concretamente a compimento. Voglio sottolineare, proprio per quel concetto che ho espresso, che si tratta di una riforma incisiva e sensibile, che merita di essere approfondita, ma non di una rivoluzione (tranquillizziamoci a questo riguardo, se qualcuno ne avesse timore), perché è stata fatta una scelta importante, giuridica

Infatti è stato sventato il pericolo che taluni facevano aleggiare che fossero compromessi i diritti di proprietà più tipici di quello che è ancora il fondamento non solo del condominio, ma dei nostri rapporti sociali e giuridici conformi e impregnati della nostra tradizione sociale, prima ancora che giuridica. Completando la mia dichiarazione di voto,

dei modi migliori - tutti cerchiamo di dare il nostro contributo - per deflazionare il contenzioso e trovare anche altre forme alternative di disciplina dei contrasti che possono insorgere. Credo di poter dire, senza tema di smentite, che il miglior modo per deflazionare il contenzioso, prevenirlo e orientare al meglio i rapporti sociali è quello di fare buone leggi leggi (leggi concretamente applicabili, non velleitarie, meno ideologiche possibile su questi terreni particolari) e tempestivamente rispondere alle mutazioni ontologiche e sociologiche della nostra società nei suoi modi d'essere e di comportarsi, in modo da dare risposta tempestiva ai fenomeni nuovi che la caratterizzano. Questi, piuttosto che inventarsi talvolta marchingegni destinati a non funzionare, sono gli strumenti migliori per prevenire il patologico contenzioso: non quello fisiologico, che talvolta può verificarsi, ma il patologico moltiplicarsi del contenzioso. Con questi sentimenti, la constatazione politica è che a questo Parlamento, al di là degli schieramenti e del gusto di polemizzare anche su ciò che polemica non richiede, può darsi atto, nei suoi vari settori, di aver svolto un buon lavoro e di avere aperto un dialogo costruttivo con i milioni di cittadini italiani che sono concretamente interessati a questo tipo di problematica. Con questa constatazione, credo positiva, mi permetto di annunciare il convinto voto favorevole del Gruppo Popolo della Libertà.

senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. è stato ivi esaminato in sede referente, e poi in sede legislativa, dalla competente Commissione della Camera ed è stato approvato all'unanimità. Esso riforma alcuni profili dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana, solidarietà italiana, (OSSI), attualmente disciplinato dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, al fine di attestare il merito di chiunque abbia specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia, sia cittadino italiano all'estero che straniero. Ricordo in proposito le perdite subite e l'importante ruolo anche della mia Regione, il Veneto, e delle Regioni del Nord Est d'Italia in occasione del secondo dopoguerra. L'OSSI è amministrato da un consiglio, composto da un presidente e quattro membri. Il presidente è il Ministro degli affari esteri che, in caso di impedimento, viene sostituito dal capo del cerimoniale del Dicastero, peraltro membro di diritto del consiglio. I restanti membri sono scelti tra funzionari della pubblica amministrazione di grado non inferiore al quinto. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio. dell'OSSI concernenti insegne, diplomi e cancelleria gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Le innovazioni recate dal disegno di legge in esame sostituiscono il riferimento ai meriti per la ricostruzione dell'Italia - ora datato - con le particolari benemerenze nella promozione di rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi. Si muta altresì la denominazione dell' OSSI in «Ordine della Stella d'Italia». Il provvedimento qualifica pertanto le onorificenze nazionali, consentendone un'equilibrata distribuzione nel contesto internazionale e ampliando la platea dei potenziali destinatari. In particolare, va ricordato l'articolo 1, che provvede alla sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, prevedendo il passaggio da tre a cinque classi di onorificenza conferenti, rispettivamente, i titoli di cavaliere di gran croce, grande ufficiale, commendatore, ufficiale e cavaliere. È prevista inoltre l'introduzione di una classe speciale che conferisce il titolo di gran croce d'onore quale riconoscimento a soggetti caduti o gravemente feriti nello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario. I criteri di conferimento e di revoca delle onorificenze, nonché le caratteristiche dell'Ordine della Stella d'Italia, sono disciplinati mediante regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Esso verrà adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e finanze. L'articolo 2 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, propongo l'approvazione da parte dell'Assemblea di tale provvedimento.

noi abbiamo iniziato il 2011 con poche ore, si potrebbe dire minuti, di lavoro d'Aula e di Commissione, molto probabilmente perché la politica italiana è distratta da altre cose che poco hanno a che fare con l'interesse dei cittadini, ma anche perché troppo spesso, sia all'inizio della legislatura che con il passare del tempo, vengono presentati disegni di legge che hanno merito e che interessano milioni di italiani ma che - magari proprio per questo - vengono accantonati o addirittura boicottati: sicuramente infatti avviano lentamente il proprio procedimento in sede di Commissione, e lì si bloccano.

decine e decine di progetti di legge e di disegni di legge che possono interessare milioni di persone, ma che invece giacciono nei cassetti delle Commissioni senza neanche avere ricevuto un parere generale relativamente ai temi di discussione degli stessi. Oggi ci troviamo a discutere, come primo o comunque tra i primi provvedimenti dell'anno, dell'adozione delle modifiche e integrazioni ad un decreto legislativo del 1948 recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana. le onorificenze e le benemerenze forse appartengono, anche dal punto di vista lessicale, agli anni in cui furono adottati, cioè immediatamente dopo la la Seconda guerra mondiale. Oggi, nel 2011, il fatto di trovarci addirittura in Aula ad occupare del tempo per discutere di modifiche ad un Ordine credo debba dare da pensare, sia nel metodo, perché, ripeto, nelle poche ore di lavoro del nostro Senato si dà priorità a questo tipo di provvedimenti, sia nel merito. Perché? All'articolo 1, comma 1, si dice che «è istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia». Immagino che ciò possa essere considerato una sorta di logica evoluzione di quanto in Italia è avvenuto due anni e mezzo fa. Sicuramente tutti voi, o quanto meno la grande maggioranza dei senatori presenti in Aula oggi, avrete votato a favore del Trattato di amicizia Italia-Libia. Sicuramente chi, a partire dall'inizio degli anni Novanta - e non c'è stata differenziazione da parte di nessun Governo, ahinoi, negli ultimi 15 anni - si è prodotto per avvicinare e consolidare i rapporti tra Italia e Libia sarà un degno candidato per ricevere questa Stella, che in qualche modo riconosce le benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e altri Paesi. Non ci si pone minimamente il problema del tipo di rapporti che il nostro Paese andrà a intrattenere o ha intrattenuto con questo tipo di Paesi,

vivano. La Libia mi pare, tranne che nelle aule parlamentari in Italia, un caso di scuola di violazione sistematica, quotidiana, dei fondamentali diritti umani. Posso fare un caso, magari meno eclatante, ma che in queste ultime due settimane ha occupato, finalmente, la stampa italiana (la peggiore in tutto il panorama democratico): quello della Tunisia. Per 25 anni il nostro Governo ha sviluppato ottimi rapporti con il regime di Ben Ali, e quindi tutti, dal 1983 ad oggi, i Presidenti del Consiglio, i Ministri degli esteri e anche le delegazioni parlamentari di amicizia (perché se ne sono susseguite negli anni) che hanno rafforzato i rapporti con la Tunisia saranno, giustamente, secondo questo disegno di legge, ottimi candidati ottimi candidati per ricevere l'Ordine della Stella. Ebbene, che cosa è successo in Tunisia lo stiamo scoprendo adesso: 25 anni di regime, magari non sanguinario e violento come quello di Gheddafi, ma altrettanto liberticida e distruttore della minima possibilità di espressione di dissenso civile, politico, sociale e, in ultima istanza, anche economico. Vogliamo fare un altro esempio? Facciamolo: la Bielorussia. Si sono tenute a metà dicembre elezioni in cui, da una parte, era stato proibito a una decina di candidati di partecipare alle elezioni, dall'altra, quando questi comunque, accondiscendendo alle prepotenze del dittatore Lukashenko, sono riusciti a partecipare, il giorno delle elezioni o all'indomani delle elezioni, quando sono state tenute manifestazioni di piazza, sei dei più noti sono stati incarcerati e con loro i giovani che li sostenevano, e a oggi non se ne ha notizia. Che cosa è successo una settimana dopo queste elezioni? Che il Ministro degli esteri della Bielorussia è venuto a Roma ed è stato ricevuto dal ministro Frattini come si confà ad un omologo, ma non è stata spesa una parola che fosse una per i candidati alternativi alla Presidenza della Repubblica che erano stati incarcerati senza motivo. Infatti, le manifestazioni temperatura di 20 gradi centigradi sotto zero, a Minsk erano tutte pacifiche e non violente e chiedevano la verifica ulteriore delle elezioni, che la comunità internazionale, colà presente, aveva dichiarato essere illegali e sicuramente non trasparenti. Non è stata spesa una parola. Vogliamo fare un altro esempio? Facciamo un altro esempio: la Corea del Nord. L'Italia da almeno 15 anni ha sviluppato un rapporto privilegiato nei confronti della Corea del Nord, tant'è vero che il penultimo ambasciatore italiano che si trovava a Pyongyang c'è stato ben nove anni. Ora, possibile che in nove anni nessuno si sia reso conto che si trattava di un regime da *gulag* veri e propri? Dubito che questo possa essere il caso, visto e considerato che in questi nove anni non soltanto non si è mai avuto un documento che in qualche modo ponesse il dubbio - mettiamola così - che in effetti il regime della famiglia di Kim Il Sung fosse quella terribile dittatura comunista - attenzione! - di estrazione tra il sovietico e il marxista-leninista, con delle sfumature confuciane, che era. Non si è saputo nulla, né tanto meno si è ipotizzata la possibilità di far comportare la nostra rappresentanza diplomatica in Corea del Nord in maniera differente. Vogliamo fare un altro esempio, e con questo concludo? La Birmania. L'Italia non solo, anche lì, è rimasta sempre presente e non è mai riuscita a spendere una parola di critica nei confronti della giunta militare che all'inizio degli anni Novanta ha cancellato le elezioni, democraticamente tenute e riconosciute dalla comunità internazionale, che fecero vincere Aung San Suu Kyi per la libertà della quale tutti poi si sono stracciati le vesti, in particolare da quando ha vinto il premio Nobel. Non si è sentita una parola, né si è mai intrapresa un'iniziativa, "stellare" per l'appunto, per interrompere i rapporti commerciali e diplomatici nei confronti della Birmania - che ha addirittura cambiato nome, nel silenzio di tutti, chiamandosi oggi Myanmar e pochi se lo ricordano, fortunatamente - ma si è mantenuta costante l'amicizia con quel Governo, e mi immagino che chi, da una parte, l'ha favorita e, dall'altra, non l'ha impedita oggi sia un ulteriore candidato per tenere sul petto la Stella dell'Ordine che vogliamo modificare.

per certi versi trovare delle giustificazioni: «È istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subìto subìto gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all'estero». Sono tre anni che il Ministero della difesa subisce dei tagli orizzontali; sono tre anni che si continua, allo stesso tempo, a rafforzare la nostra presenza sui teatri internazionali, sia che si tratti di missioni delle Nazioni Unite, sia che si tratti di missioni dell'Unione europea. Oggi che cosa si fa?

e velocità all'adozione di disegni di legge totalmente inutili, che non fanno tesoro dei principi della nostra Costituzione, né tantomeno dell'obbligo che l'Italia dovrebbe rispettare di proteggere e promuovere i diritti umani nel mondo, perché qui si parla soltanto di amicizia tra i Governi, un terzo dei Governi nel pianeta non è a legittimazione democratica: quindi, quanti più amici tra i peggiori mi faccio, quante più stellette d'onore (o comunque si vada a chiamare questo nuovo ordine) posso mettere alla mia giacchetta. Noi diamo grande importanza all'adozione di questo tipo di

visto e considerato quello che succede. Infatti, non si tratta di mercificazione del corpo, ma soltanto di uno scambio: io do delle prestazioni, in questo caso sessuali, vengo pagato e il problema si dovrebbe

Per contro, vi sono dei costi per il cittadino: tra i 3.000 e i 13.000 euro dalla separazione al divorzio. Attualmente, i tempi per il divorzio sono più o meno di due anni

che giacciono nelle Commissioni competenti che potrebbero portare un risparmio notevole alle casse dello Stato. Ripeto: 842 euro è il costo per ogni separazione e 815 il costo per ogni divorzio. I divorzi sono 178 ogni 1.000 matrimoni (un numero

parziali rispetto alle tematiche generali da lui evocate. Ritengo si tratti di uno strumento utile per

di uno strumento di adeguamento di norme esistenti da tempo immemorabile che devono trovare adattamento alle nuove situazioni.

in dedica e solidarietà a tutte le vittime dell'uranio impoverito, perché si corre il rischio che, dopo dieci anni di processi, si vedano insignite esclusivamente della Stella, piuttosto che ricevere giustizia e una riparazione,

e che coloro che sviluppano l'amicizia tra l'Italia e un altro Paese debbano avere titolo alle onorificenze ufficiali della Repubblica. Abbiamo un Ordine al merito della Repubblica italiana: si insigniscano le persone che hanno benemerenze in questo campo dell'Ordine ufficiale della nostra Repubblica: creare un Ordine separato significa ghettizzare le persone che avranno quell'onorificenza, svalutare

Ilrelatore, senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

nuove norme in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Si tratta, quindi, di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali

con contratto regolato dalla legge dello Stato di residenza. Si tratta di permettere a questi lavoratori di partecipare alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.

che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alla elezione delle rappresentanze RSU. Questo vuol dire che viene escluso da questo diritto il personale in servizio presso le sedi diplomatiche consolari e presso gli istituti italiani di cultura all'estero, il quale è assunto sulla base di contratti regolati dalla legge locale.

un comma 3-*bis* per la partecipazione alla rappresentanza sindacale unitaria; inoltre, garantisce la partecipazione del personale

La prima è che l'attuazione del disegno di legge non abbia costi aggiuntivi, cioè che avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

a doverci regolare fra due opposte o complementari situazioni. La prima è di tutelare comunque i regolamenti già consolidati del personale del Ministero con contratto a tempo indeterminato.

potremmo identificare una pausa prima di approvare il testo. Non intendo un rinvio in Commissione *sic et simpliciter*, ma un rinvio in Commissione con la contemporanea costituzione di un gruppo di lavoro ristretto,

perché, ci dice il relatore, i sindacati confederali del Ministero degli affari esteri si oppongono, e sono riusciti in ventiquattrore a far rovesciare al Governo la sua posizione e a bloccare questa maggioranza.

di sindacati confederali del Ministero degli affari esteri, che io considero delle vere e proprie corporazioni. A mia conoscenza, caro relatore, la CGIL nazionale chiedeva di approvare questo disegno di legge: dunque opportuno chiarire qual è la posizione del sindacato confederale e della rappresentanza delle corporazioni del Ministero degli affari esteri. Vedete, questo problema mette in evidenza le difficoltà che abbiamo con il Ministero degli affari esteri. e dovremmo iniziare a lavorarci prossimamente - un'indagine conoscitiva sul funzionamento del Ministero degli affari esteri, in particolare sull'utilizzo delle risorse umane ed economiche nella rete consolare.

I parlamentari di tutte le parti politiche hanno segnalato al Ministero degli affari esteri un problema estremamente serio nel secondo consolato italiano nel mondo. Il Ministro degli affari esteri, parlando di questo problema, ha dovuto riconoscere che è impotente ad agire nei confronti di un reggente consolare.

del relatore, e io mi permetto di consigliargli ancora una breve riflessione al ritirare la proposta di rinvio in Commissione e di far votare questo disegno di legge. Questa è la risposta che aspettano persone che lavorano per l'Italia e che non stanno difendendo loro privilegi, come quelli che ben conosciamo al Ministero degli affari esteri.

Signora Presidente, vorrei fare una breve considerazione a sostegno della posizione particolarmente saggia e prudente esposta dal relatore.

all'elezione della rappresentanza sindacale unitaria lavoratori i quali non sono espressione del contratto come invece le RSU che dovrebbero votare. Sarebbe come se in un'azienda un'azienda ad eleggere i rappresentanti sindacali unitari fossero chiamati i dipendenti di una cooperativa. Il che non nega, evidentemente, che i lavoratori di quella cooperativa svolgano un ruolo importante in quel circuito produttivo e organizzativo, ma hanno un'alterità contrattuale superarla, chiamandoli ad una contaminatoria commistione in termini di riferimento della rappresentanza, è un principio - guardo anche i colleghi della Commissione lavoro - particolarmente insidioso. Credo, che la proposta del relatore possa consentire alla Commissione lavoro una valutazione più accurata di un profilo che, se riverberato su altre dimensioni, potrebbe essere non privo di rischi. *(Applausi

che ha richiesto un rinvio in Commissione, rinvio che può trasformarsi in ritorno in tempi opportunamente brevi. Signora Presidente, siamo rimasti, oltre che meravigliati, anche sconcertati dalla presa di posizione del relatore.

che va a tutelare, e non a penalizzare. Oggi si è di nuovo parlato della penalizzazione addirittura dei contrattisti.

Senatore Bettamio, lei ha sentito il dibattito e la reazione dei vari Gruppi. La richiesta mi pare sia in

Parlamento, è di evitare che l'esclusione dei dipendenti del Ministero che lavorino *in loco* con un contratto diverso da quello dei loro colleghi

nel modo più efficace possibile, in modo tale da non contrastare né le rappresentanze sindacali, né i diritti di quelli che lavorano all'estero o nel nostro Paese. La logica della proposta è di ritornare in Commissione e costituire un gruppo di riflessione, coordinato dai

Presidente, penso che un breve rinvio in Commissione per un approfondimento particolare

anche per dialogare con queste corporazioni, non sia sbagliata: è un atto di saggezza, se lo lasci dire da chi ha qualche anno in più.

Scotti, è certo che il mondo del lavoro è diviso in gruppi che premono da una parte o dall'altra, però il compito della politica sarebbe quello di capire qual è l'interesse generale. Come ha messo in rilievo il collega senatore Micheloni, l'interesse generale del Paese qui sta dalla parte di chi vuole cambiare, naturalmente cercando il consenso: non si vuole cambiare contro il personale del Ministero degli affari però del tutto evidente, cifre alla mano, come ricordava il collega Micheloni, che tutti i Paesi europei ormai hanno nella loro rete consolare, in particolare in Europa, una prevalenza di personale *in loco* piuttosto che di personale inviato da Roma. Roma. Sappiamo che tutti gli anni abbiamo a che fare con restrizioni del bilancio del Ministero degli affari esteri. Allora, quanto a lungo potremo andare avanti con una struttura del bilancio come questa?

avete chiesto il voto in nome del cambiamento dell'Italia: se vi fermate di fronte a un gruppo di questo genere, è evidente che tale promessa non può essere mantenuta. È con questo spirito che voteremo a favore della proposta di